grazie a tutta

del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 361-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

la Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, aveva trovato un punto di equilibrio, tant'è vero che il Gruppo di Forza Italia votò a favore del provvedimento, come pure votò a favore in occasione dell'approvazione nel Senato della Repubblica nel maggio 2016. Successivamente il provvedimento fu inviato alla Camera, dove abbastanza inspiegabilmente, dopo il duro lavoro fatto dal Senato, giacque sostanzialmente per circa un anno e mezzo,

non usò il metodo della condivisione e della ricerca di equilibrio e, soprattutto in alcuni parti del provvedimento,

che, quando il provvedimento ritornò al Senato, in Commissione sanità chiedemmo delle audizioni per conoscere, direttamente dagli interessati,

la loro assoluta contrarietà nel merito della questione. Questi sono i motivi per i quali il Gruppo di Forza Italia manifesta condivisione per la parte che aveva già condiviso, ma assoluta contrarietà per quanto fatto dalla Camera, soprattutto per gli articoli 4 e 6, sugli ordini e la razionalizzazione delle professioni sanitarie, perché, di fatto,

di questa legislatura, dire: prendere o lasciare. Abbiamo notevoli perplessità su questo provvedimento, considerato anche il fatto che il nostro Gruppo parlamentare alla Camera ha votato contro il provvedimento per le motivazioni che ho appena illustrato. *(Applausi dal

Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il disegno di legge che viene oggi presentato e dibattuto in Aula riporta norme che si riferiscono ad aree tematiche diverse ma collegate e legate da un filo rosso conduttore. Diversi gli obiettivi: risistemare la riforma della normativa sulla sperimentazione clinica, coordinare i Comitati etici

ancorché ultra ventennale, che finalmente potrà trovare un formale e giuridicamente certo riconoscimento attraverso un riordino che coinvolge tutte le professioni sanitarie superando finalmente alcune criticità, alcuni vuoti, che le leggi attuali non possono colmare e che, senza l'intervento di questo disegno di legge, non si sarebbero potute superare. n. 1324-B ridefinisce le pene per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria al fine di proteggere e tutelare i cittadini da lestofanti, maghi e fattucchieri; indica un chiaro percorso per quanto attiene la formazione medica specialistica e di formazione dei medici extracomunitari; riporta alcune disposizioni per il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e norma la dirigenza sanitaria del ministero della salute. Un disegno di legge, dunque, importante e complesso che commenterò per una sua attesissima parte: quella che tratta il tema del riordino delle professioni sanitarie. In questo momento, signor Presidente e onorevoli Senatrici e Senatori migliaia di professionisti ci stanno guardando ed ascoltando, nell'attesa del voto definitivo che sancirà un attesissimo traguardo storico e che vorrebbero, auspicherebbero bipartisan. Dopo un lungo lasso temporale ed un impegno più che biennale delle due Camere, si è giunti, da una parte, al riordino ed alla novellazione delle norme grazie a tutta grazie a tutta

possono compiutamente e finalmente essere definite come un ulteriore passo in avanti non tanto e non solo per l'oltre un milione di professionisti sanitari operativi nel nostro Paese, quanto per i cittadini italiani ed europei che fruiscono delle loro prestazioni professionali La tanto attesa riforma ordinistica in sanità lascia alle spalle, e finalmente, un percorso tortuoso e accidentato fatto di "*stop and go*", di speranze e acerbe delusioni rese ancora più incomprensibili per l'acclarata evidenza di quanto il previgente e attuale impianto ordinistico avesse bisogno di un'ampia

grazie a tutta grazie a tutta di radiologia medica le professioni sanitarie al momento prive di Albo dimostrando la capacità di effettuare una scelta che ha subordinato l'interesse particolare a quello generale. E, in ultimo e permettete, un virtuale braccio alle tante donne e ai tanti uomini delle professioni sanitarie tutte

Dichiara altresì improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, la proposta 15.0.200 in materia di età di quiescenza dei professori ordinari, in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge che reca invece disposizioni in materia sanitaria.

di evitare il disallineamento tra l'elezione degli ordini e l'operatività del disegno di legge in oggetto, posto che la legge entrerebbe in funzione a fine gennaio e comunque, per essere attuativa, avrebbe necessità di provvedimenti governativi anche di natura regolamentare per cui andrebbe a contrastare con le elezioni degli ordini già effettuate, con quelle che sono in fase di effettuazione

il parere favorevole

Avremo così più trasparenza negli ordini professionali, con l'inserimento del *turnover* e della parità di genere, nonché di pene più severe per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Si riconoscono due nuovi ordini professionali, quello degli osteopati e quello dei chiropratici, e poi avremo anche più tutele per i pazienti ricoverati nelle strutture sia pubbliche che private, introducendo pene più severe per i reati contro la persona. Con il mio Gruppo Italia dei Valori voteremo sicuramente di sì a questo disegno di legge e ritengo così di aver fatto il mio dovere di legislatore. Voglio però ricordare che il rapporto medico-paziente non è fatto solo di norme, anche se ben scritte: alla base di questo dobbiamo pensare sempre che ci

alcuni passi e ringrazio tutta la Commissione sanità, che molte volte mi ha anche sopportato, oltre che supportato, ritengo però fondamentale far comprendere che abbiamo portato quasi a un metro dall'arrivo molti disegni di legge che andavano in questa direzione, per cercare più empatia e più fiducia nel rapporto medico-paziente.

imporre un obbligo sanitario in questo modo, senza un reale bisogno, abbia creato soltanto la diffidenza di molti pazienti verso i medici e soprattutto la riduzione di quell'empatia che considero

per essere approvato in seconda lettura, senza possibilità emendativa, nonostante sia stato ampiamente modificato rispetto alla versione uscita dal Senato. Questo disegno di legge, mi verrebbe da dire, è un vero e proprio «trenino»

con la finalità di individuare con certezza i comitati etici territoriali, cui sono stati affiancati comitati etici a valenza nazionale; argomento certo condivisibile ed importante sul quale però noi al Senato non abbiamo potuto incidere. aggiunto l'articolo 3, concernente l'applicazione e la diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale. Hanno anche aggiunto l'articolo 5, che istituisce le nuove figure professionali sociosanitarie; figure professionali certamente necessarie, ma alcuni profili hanno due percorsi culturali diversi. Nell'ambito della figura dell'educatore professionale, ad esempio, si possono avere due percorsi universitari diversi: i corsi di laurea delle classi L-19 Scienze dell'educazione e della formazione e L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione. Pertanto sarebbe necessario un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra le facoltà di Scienze della formazione e le facoltà di Medicina, per unificare i due percorsi e non penalizzare nessuno. aggiunto l'articolo 6 che va a riscrivere l'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, articolo che permetteva di individuare ed ora anche di istituire le nuove professioni sanitarie. Perché non è stato fatto funzionare per tutte? Perché creare figli e figliastri, qual è la necessità di istituire alcune professioni sanitarie (certamente legittime) come l'osteopata e il chiropratico e non altre, come ad esempio il laureato in scienze motorie? Hanno quindi aggiunto l'articolo 11, che va a modificare la legge 8 marzo 2017, n. 24. Sì, cari cittadini, avete capito bene, si mette mano, dopo nove mesi dall'approvazione, alla legge sulla responsabilità professionale,

Avete visto che tagliando di revisione? Pensate se aveste comprato un'automobile e dopo nove mesi foste obbligati a revisionarla completamente, cosa pensereste dei progettisti di tale veicolo?

recante disposizioni particolari per i medici extracomunitari, nel decreto legislativo n. 286 del 1998. Mi fa davvero molto piacere che possiamo insegnare per due anni ai professionisti in attesa dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso, ma non posso non rilevare però come molti nostri laureati lascino l'Italia per mancanza di possibilità di inserimento. Forse un giusto equilibrio sarebbe necessario. un provvedimento di 18 articoli, arriva al Senato con 6 articoli nuovi di zecca più altri commi qua e là, che non possono essere discussi perché il provvedimento è blindato. Il capolavoro comunque resta in assoluto l'articolo 17, il marchettone dell'emendamento Polverini del 2013. L'ho già spiegato ieri nella discussione generale e non lo riprendo, però è fenomenale, che un articolo bocciato per ben tre volte, ma caparbiamente ripresentato con un'incredibile faccia tosta, a turno dai vari schieramenti PDL e "PD meno L" - mi verrebbe da dire «chi la dura la vince» - viene finalmente approvato dopo quattro anni dal suo esordio. L'articolo 1, che prevede la delega al Governo per la sperimentazione clinica, ci appare molto debole: come garantire l'assenza di conflitto di interesse - comma 2, lettera *d)* - e come diffondere i risultati positivi e negativi delle sperimentazioni precliniche, nonché di tutti i *trial* clinici, indipendentemente dal loro esito? Inoltre, i dati inclusi nel rapporto su uno studio clinico non dovrebbero essere considerati informazioni commerciali, anche se di carattere riservato. È di questi giorni la pubblicazione di libri sul conflitto di interessi di rappresentanti della sanità pubblica: non dite nulla? Quale credibilità ritenete di acquisire sui cittadini? Li disorientate e poi vi lamentate se vi contestano; è una vera vergogna. Termino il mio intervento commentando l'articolo 4, sul riordino della disciplina delle professioni sanitarie, articolo che istituisce albi e ordini professionali con struttura organizzativa rigida, voluta per lo più dagli organi dirigenziali che non dalla base. La prova provata di quel che dico si rende evidente nella gestione degli ordini e dei collegi cosiddetti storici: alle votazioni dei rinnovi delle cariche la percentuale dei votanti è spesso sotto il 10 Forse si doveva partire da questa analisi per cercare di capire quello che la base ovvero i professionisti chiedono e di cui hanno bisogno. Io sono iscritto all'Ordine dei medici e non se sento né la necessità, né il bisogno. Andava ricercata una maggior partecipazione e responsabilizzazione, dando il diritto di poter contare: se in una votazione non si arriva alla maggioranza degli aventi diritto, come in un *referendum*, l'ordine provinciale sparisce e viene assorbito da quello regionale. Invece, si è fatto esattamente l'opposto: si dà potere al rappresentante legale, tanto poi pagano gli iscritti, spesso alla canna del gas, precari,

manca una vera spinta innovativa. Si tratta di un testo che, fin dalla prima versione, non introduce un'effettiva modernizzazione del sistema ordinistico. Il disegno di legge Lorenzin, nato infatti dall'esigenza di una modernizzazione delle norme istitutive degli ordini e dei collegi professionali risalenti a più di sessant'anni fa, già dalla prima versione appariva privo di quella spinta innovativa capace di incidere sul vigente sistema ordinistico per superare quegli aspetti non più rispondenti al mutato mutato contesto politico, sociale ed economico in cui operano le professioni sanitarie. Si tratta di un impianto normativo che non affronta il cuore delle questioni, ma che interviene su specifici punti del testo del 1946 senza proporre nel suo complesso una disciplina effettivamente nuova, moderna ed efficace. Il testo approvato dalla Camera è una riscrittura del testo del 1946 che demolisce, di fatto, l'autonomia ordinistica; un testo che in qualche modo è decisamente negativo sull'autonomia degli ordini, che è peraltro un requisito caratteristico di tali enti e delle specifiche funzioni che questi svolgono in relazione

di fatto lasceremo questa legislatura con un *pot-pourri* del tutto sospeso. Quali garanzie per il futuro? Sicuramente nessuna, perché è tutto molto vago. La modificazione del *quorum* necessario per la validità dell'assemblea elettorale e la previsione di tre convocazioni per quanto riguarda gli ordini, nonché l'introduzione del voto per via telematica, renderà tutto più farraginoso e lungo, con complicazioni operative delle quali proprio non si comprende la *ratio*, visto che, come diceva prima il collega Gaetti, già ora la situazione è abbastanza complicata. anche di altri aspetti, ma vorrei puntualizzare un concetto che deve essere chiaro. Diciamo che le professioni sanitarie sono ancora una giungla, perché alcune preparazioni universitarie vengono equiparate ad altri grazie a tutta

che garantiscono e certificano l'unicità dell'azione. È lo Stato che si fa garante di quelle professioni che hanno un elevato grado di responsabilità. Non possiamo fare un albo per ogni professione perché, di fatto, a quel punto ne annulleremmo il valore di garanzia a tutela del cittadino, del paziente, e non della professione stessa. Certe professioni non necessitano di un albo. Partiamo quindi dai profili di formazione; partiamo dalla professionalità e dalle responsabilità. La responsabilità, di fatto, a chi va poi? Facciamo tutti questi albi e diamo la responsabilità o la responsabilità

La cosa più assurda, però, è la schizofrenia di trovare, ad esempio, una discrepanza tra gli ordini nazionali e quelli provinciali che, quando mancano i numeri, pur di salvare

per creare ulteriore disordine. Quello che bisognava fare, quindi, era incidere sulla formazione, cosa che non piace perché costa fatica. Ebbene sì, le cariche,

Dico anche un'altra cosa. Ma quando si prende a modello l'estero, vogliamo piuttosto dire che noi, ad oggi, con la formazione che abbiamo avuto finora,

tradizionale classico era valido. E, a garanzia, ci mettiamo meno soldi? Allora adesso cosa facciamo: derubrichiamo e diminuiamo la formazione e la qualità? Poi, però, voglio vedervi quando, come pazienti, finirete di quello che ha fatto un corso di cinque giorni, cinque settimane o cinque mesi, a differenza di chi ha fatto un percorso di anni e anni (e non bastano mai!). Andiamo ad altri punti. Il limite di mandati consecutivi per quanto riguarda gli ordini merita un'attenta considerazione, perché questi vanno ad impedire che gli incarichi elettivi possano essere ricoperti per più di due mandati consecutivi, trattandosi di interventi che ristrutturano l'attuale assetto Un eccessivo e forzato avvicendamento delle cariche di vertice rischia infatti di minare la stabilità di tali enti, nonché di impedire la programmazione di politica professionale e, conseguentemente, la realizzazione degli stessi. Al contrario di quanto chiarito per i consigli direttivi degli ordini provinciali, per i comitati centrali continua ad essere previsto, in caso di scioglimento, che sia nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, grazie a tutta

La modifica apportata dall'Aula appare in ogni caso inadeguata, in quanto continua a permanere un dubbio interpretativo circa la possibilità per un ordine di non recepire il codice deontologico approvato dalla federazione nazionale. Appare dunque fortemente contraddittorio richiedere la maggioranza di due terzi per l'approvazione del codice deontologico e poi non prevedere la sua obbligatorietà su tutto il territorio nazionale. Non è corretto neppure il richiamo al comma 18 nel comma 1 dell'articolo 4, capoverso «Art. 8», comma 19, che appare errato in quanto in tal modo sembrerebbe che contro tutti i provvedimenti, anche non disciplinari, assunti dai comitati centrali si debba ricorrere alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. È previsto inoltre che fino all'adozione dei nuovi regolamenti governativi trovino applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto In proposito si evidenzia che l'utilizzo di tale locuzione crea numerose criticità interpretative che potrebbero dar luogo a contenziosi, in quanto è solo la magistratura ad avere la competenza a valutare l'eventuale abrogazione tacita per incompatibilità. Una situazione di tal genere si sta già riscontrando nell'ambito dell'applicazione della normativa sulla gestione societaria delle farmacie, come modificata da ultimo dalla legge n. 124 del 2017, che contiene un'espressione identica in materia di disciplina sull'incompatibilità per i soci e che sta creando notevoli difficoltà di interpretazione. È pertanto preferibile prevedere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della normativa che disciplina gli ordini Si segnala inoltre che, mentre per le federazioni nazionali i relativi regolamenti di organizzazione restano efficaci fino all'adozione degli statuti, per gli ordini provinciali non è stabilita la medesima previsione; per questi ultimi è dunque necessario che sia previsto che, fino all'adozione dello statuto da parte della relativa federazione nazionale, continuino ad applicarsi i regolamenti interni vigenti. Come dicevo, c'è una gran confusione:

previsione che consente a tante altre categorie operanti nei vari ruoli sanitari di potersi organizzare all'interno di un ordine professionale. Mi permetto solo di dire che ovviamente siamo più che favorevoli all'approvazione del provvedimento e salto i ringraziamenti di rito per dire che probabilmente è sfuggito Gli ordini professionali non avranno più una funzione ausiliaria per la pubblica amministrazione ma sussidiaria; che non solo terminologicamente, ma dal punto di vista del significato del diritto amministrativo non saranno più solo di ausilio, ma saranno delegati loro dei compiti decisionali che sono propri dell'ordinamento di sussidiarietà. Ciò significa valorizzare la funzione del organi professionali, che non saranno più chiamati a fare i cerberi e a valutare i comportamenti difformi rispetto all'ortodossia deontologica, ma potranno, secondo il principio di sussidiarietà, proporre miglioramenti nell'ambito della stessa professione.

la sanità ha una particolare configurazione che non hanno altre attività. Nelle altre attività della pubblica amministrazione si può anche decidere di non disciplinare, di non controllare e di non vigilare e ciò potrebbe anche portare un risparmio in agricoltura, nei lavori pubblici e in qualche altro ambito di intervento della pubblica amministrazione. In sanità invece è l'esatto contrario: ogniqualvolta non si disciplina e non si adegua la normativa alle mutate esigenze sanitarie, si producono non solo disservizi e carenza di assistenza ma anche un aumento del debito sanitario. Quindi ben venga ogni provvedimento che vada nella direzione di una più moderna disciplina e di una maggiore dinamicità dell'ambito normativo, all'interno del quale i singoli professionisti si vanno a muovere. Ho letto sui giornali che c'è stata qualche doglianza, ma non voglio fare polemiche con nessuno. Noi siamo ormai una società a democrazia avanzata. Capisco che ci sono ordini più autorevoli, perché più più accorsati, come quello dei medici, dei farmacisti e degli avvocati. Credo però che con l'evoluzione dei tempi - che non sta modificando i rapporti di forza, perché l'autorevolezza viene dalla funzione che si svolge e non dal numero degli iscritti iscritti - la sanità italiana più che di guerre intestine abbia bisogno di un principio di concordia, perché alla fine la *mission*

sempre la somma di tanti piccoli interventi, spesso destinati a tacitare alcune richieste, ma senza una visione complessiva che li ricollegasse. Dei 26 articoli iniziali, 16 sono stati subito stralciati quando la Commissione sanità del Senato ha cominciato a lavorare sul testo, per cercare di concentrarsi su ciò che era più importante. Questo provvedimento arriva oggi ad essere approvato, nonostante il provvedimento originale che ci è arrivato dal Governo, grazie al lavoro delle due Commissioni competenti di Camera e Senato, che voglio qui ringraziare espressamente. affronta alcuni temi che sono assolutamente importanti, anche se su alcuni aspetti il modo con il quale li affronta possono non essere condivisi. Mi soffermo su poche questioni. L'articolo 1 riguarda le sperimentazioni cliniche, le sperimentazioni cliniche, che necessitano da tempo - come sappiamo - di un riordino culturale, prima che legislativo. Questo riordino è estremamente importante. Come abbiamo detto in Aula e in Commissione, la proposta del Governo era estremamente carente sul tema, perché tutto il mondo scientifico sa che sulle sperimentazioni cliniche ciò che manca in modo particolare è una definizione dei principi etici per la ricerca clinica. Di questo il provvedimento che ci era arrivato non parlava affatto.

di Helsinki proprio sulle questioni etiche che è del 1964 e che è stata inserita dopo. Per fortuna nel frattempo è arrivato un regolamento dell'Unione Europea, al quale abbiamo potuto fare riferimento, e abbiamo potuto scrivere principi volti a tutelare l'indipendenza delle sperimentazioni e l'assenza di conflitti di interesse sia tra i ricercatori, che tra i responsabili e i valutatori. valutatori. È una questione estremamente importante, come il Governo sa. Il Governo sicuramente conosce la differenza tra una condizione di conflitto di interesse e un comportamento di conflitto d'interesse. Aspettiamo ancora la risposta ad un'interrogazione a mia prima firma, firmata anche da molti altri senatori, sui conflitti di interesse di importanti responsabili di enti vigilati dal Ministero della salute sul tema delle vaccinazioni,

Ci sarebbe stato bisogno di lavorare di più sulla ricerca senza scopo di lucro: l'abbiamo introdotta noi, prima, in Commissione igiene e sanità e poi è stata ulteriormente migliorata alla Camera dei deputati, perché tutta la ricerca e la sperimentazione clinica, svolta dagli studi

dell'università sia soggetto alle stesse regole, se non ce n'è bisogno. Abbiamo cercato di introdurre questo principio, altrimenti ciò vuol dire che si vuole fare terra bruciata intorno alle multinazionali, affinché la ricerca senza scopo di lucro non abbia futuro. Su questo abbiamo lavorato anche in Commissione, perché qualche volta il Governo ha dimenticato la ricerca indipendente in sanità. Non mi soffermo ulteriormente su questo aspetto, perché il rispetto degli *standard* internazionali di etica nella ricerca medica è stato ben precisato nella legge, che è una legge delega e ha dunque tanti principi tanti punti, e ci auguriamo che i provvedimenti che dovranno essere adottati siano coerenti con quei principi. Mi soffermo ancora su un altro punto: il riordino degli ordini - scusate il bisticcio di parole - estremamente importante. Gli ordini sono enti pubblici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare interessi pubblici e quindi hanno un ruolo fondamentale. Non ci dobbiamo stupire, perché negli anni hanno svolto dei ruoli un po' diversi da quelli che la legge attribuiva loro ‑ anche la vecchia legge ‑ sostituendosi spesso alle *lobby* o ai sindacati. Ora ci auguriamo che questa nuova versione, questa nuova disciplina degli ordini possa far nascere una stagione nuova; non solo perché gli ordini sono estesi a tutte le professioni sanitarie - cosa che ci induce con decisione a valutare positivamente il provvedimento in esame, perché "o tutti, o nessuno" - ma soprattutto perché fissa dei paletti molto chiari, che forse agli ordini più storici possono dare fastidio, perché modificano un pochino

di assistenza (LEA) e qui vorrei rivolgermi al Governo e mi dispiace non ci sia il Ministro competente. È stato stralciato giustamente, perché nel frattempo i LEA sono stati approvati, ma essi sono fermi al palo, sono fermi al palo, perché, salvo pochissimi elementi che potevano essere attuati senza provvedimenti ulteriori del Governo, la gran parte - i quattro quinti - di quel provvedimento sui LEA, che tutti noi abbiamo approvato con grande entusiasmo, è ferma, perché i nuovi tariffari di tutte le

resterà scritto sulla sabbia. Infine mi permetto di dire che sono molto felice che si possa affrontare il tema del personale medico del Ministero della salute e che si possa risolvere un annoso problema. Anche in questo caso, però, mi dispiace che tutto quello che abbiamo fatto sul personale che ha a che vedere con il settore sanitario, riguarda piccoli elementi, piccole questioni che riguardano un pugnetto di persone, mentre abbiamo completamente trascurato il tema della valorizzazione del personale, del riconoscimento del lavoro che il personale sanitario fa nonostante le restrizioni continue e nonostante le difficoltà organizzative e nonostante le continue richieste di riduzione del personale. Abbiamo perso Abbiamo perso quasi tre miliardi di spesa sul personale. Non è pensabile che un settore ad alta intensità di lavoro continui ad essere continui ad essere trattato come un settore in cui il personale è un dettaglio salvo quelli del Ministero, dell'AIFA, dell'Istituto superiore di sanità e degli IRCSS. È importante che si risolvano i problemi del personale di quegli istituti, ma bisogna guardare al personale che opera tutti i giorni davanti ai cittadini. Detto questo, siccome il provvedimento consente di fare un passo in avanti sulle sperimentazioni cliniche, sugli ordini e su altri temi, il mio Gruppo dichiara voto favorevole. Signor Presidente, accoglierò la sua sollecitazione e sarò brevissimo. Voglio dire semplicemente che questo disegno di legge, che ha avuto una gestazione lunghissima, affronta due argomenti enormi che sono, appunto, il riassetto della sperimentazione clinica e il riordino delle professioni il primo punto, naturalmente attraverso una legge delega e quindi in attesa del lavoro del Ministero per i decreti attuativi,

anche in questo caso credo che il riordino degli ordini e la nascita di nuovi ordini non possa che inserirsi nell'ottica di una valorizzazione dei professionisti della sanità. Certo, qualcuno si è lamentato, qualcuno invece è contento. Io credo che sia un passo avanti per ridare ridare vigore alle associazioni ordinistiche. C'è stata un po' di polemica sugli osteopati e i chiropratici. Io credo che, invece, questa sia l'occasione per determinare una maggiore chiarezza su due professioni sanitarie alle quali milioni di cittadini si rivolgono. Quindi, per concludere, credo che il combinato disposto della legge sulla responsabilità civile dei sanitari e questo

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, quando il 24 maggio 2016 votammo qui in Aula questo provvedimento in prima lettura, a seguito di un dibattito molto puntuale e preciso e direi anche ricco, nell'illustrazione degli emendamenti che furono approvati, si consolidò un convincimento che vide molte forze politiche, di maggioranza e di opposizione, condividerne l'impostazione, la *ratio*. Certo, si era convinti sin da allora che purtroppo il meglio è nemico del bene e quindi, diciamo che ci si convinse che quello era un provvedimento che poteva ottenere il voto positivo. E così fu.

- è accaduto quello che non dovrebbe accadere con riferimento al lavoro che devono svolgere i due rami del Parlamento, nel senso che

dare maggiore forza, coerenza ed applicabilità alla norma che s'intende approvare. Così purtroppo non è stato e mi dispiace dire che non è stato per motivi attinenti alle contese interne alle forze di maggioranza che sostengono questo Governo. Signora Ministro, non è il momento di polemizzare, il Presidente ci invita a tenere i tempi stretti, ma è sufficiente dare una lettura degli interventi alla Camera per comprendere che molti dei problemi si sono sviluppati in casa PD

non lo volesse, questo provvedimento, ovvero che il Partito Democratico non fosse totalmente allineato, almeno in quell'altro ramo del Parlamento, sull'approvazione di questo provvedimento. Qui

in Aula, nella consapevolezza che esso contiene dei punti importanti - voglio dirlo con chiarezza - molti dei quali sono figli di provvedimenti legislativi provenienti dalla precedente legislatura e targati centrodestra: il tema della sperimentazione clinica, con la necessaria armonizzazione delle norme in una logica europea, che talvolta ci vede fanalino di coda, i passi in avanti sul versante della trasparenza delle modalità di svolgimento dell'attività di sperimentazione clinica, il rigore, la terzietà, l'indipendenza, le attività che ancora di più e meglio abbiamo disciplinato con riferimento ai comitati etici, la medicina di genere sono tutti elementi che sono assolutamente da considerarsi molto convincenti. Così come l'introduzione del parto indolore nei la previsione di sanzioni ancora più severe per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, la disciplina di alcune professioni *borderline* che avevano necessità di una regolamentazione tutti aspetti che indubbiamente avevano conferito e conferiscono ancora, tutto sommato, a questo provvedimento una validità. Da ultimo, c'è il tema rilevante della riforma degli ordini, ordini, che può essere definito una sorta di telenovela, perché si trascina, tra luci e ombre, nelle Aule del Parlamento, tra chi è favorevole agli ordini e chi gli ordini ritiene che siano residui residui arcaici di un'epoca passata e che non servano a nulla. Noi crediamo che gli ordini servano, che per farli servire di più e meglio nella loro funzione pubblicistica essi devono evidentemente essere ammodernati, perché le fonti legislative e regolamentari di riferimento risalgono a settant' anni fa. Così si tentò di fare, nel 2006, con la legge n. 43 che delegava il Governo ad adottare specifiche disposizioni anche per

Grazie. viceversa, sarebbero state affidate all'ambiguità ed al *vulnus* legislativo, con conseguenti ricadute negative anche per quanto riguarda gli spazi lasciati a impostori e abusivi. Purtroppo poi la fine della XIV legislatura fece decadere la delega e non se ne fece più niente. Nella scorsa legislatura,

per una serie di motivi, ritornò in Commissione, la legislatura finì e non se ne fece niente. riorganizzazione e del riammodernamento degli ordini, nonché del riconoscimento di nuovi ordini sanitari, credo che questa volta non possiamo fare un passo indietro. Non possiamo farlo, perché tradiremmo le aspettative di oltre un milione di persone, un milione di professionisti che servono il Paese su un versante particolarmente delicato. Penso ai tecnici del laboratorio biomedico, agli igienisti dentali, ai tecnici della prevenzione e della riabilitazione, agli infermieri che oggi ottengono l'ordine, essendo costituiti in collegio; penso ai tecnici di radiologia medica. un passo in avanti che serve al Paese, non a gratificare le aspettative di quelle che molto spesso vengono impropriamente considerate *lobby*. Serve al Paese per dare maggiore certezza e garanzia di efficacia e di efficienza alla qualità delle prestazioni professionali e all'attività pubblicistica che lì si deve realizzare. dovesse fare una valutazione sulla qualità della produzione legislativa comparata fra Camera e Senato, credo che il Senato sarebbe promosso a pieni voti, mentre la Camera purtroppo no, perché lì si sono pasticciate un po' le cose. Proprio sull'articolo relativo agli ordini si sono commessi gravi errori, che non tengono conto delle asimmetrie relative alle procedure elettorali per gli ordini a livello provinciale Non tengono conto del codice deontologico che, così come disciplinato nella norma modificata, potrebbe essere disapplicato in alcuni ambiti del territorio, privando in tal modo un ordine del proprio codice etico e morale di comportamento, che deve necessariamente avere una vigenza a livello nazionale. Lo stesso vale per i regolamenti interni vigenti e la loro compatibilità Non so, signora Ministro, se questo provvedimento può determinare punti di caduta, ma spero che l'ordine del giorno che è stato approvato serva a dare una risposta puntuale e precisa. Confido

dinanzi a un'incomprensibile miscela di norme poco riuscite, al posto e in sostituzione di quello - l'unica - che sarebbe stato necessario adottare a tre mesi dalla fine della legislatura, cioè un vero intervento a sostegno della sanità pubblica. Invece, ci siamo trovati dinanzi ad aggiustamenti per parti separate e frammentarie, senza un'idea di sviluppo del sistema sanitario e di rafforzamento complessivo della sanità pubblica. Il voto di oggi è quasi una beffa, perché proprio oggi si approva alla Camera dei deputati il disegno di legge di bilancio. Quella legge di bilancio che conferma tagli alla sanità; quella legge di bilancio che conferma che non si fa un investimento serio sul personale sanitario, da sempre non solo poco valorizzato, ma con stipendi bassissimi; una legge di bilancio che non rafforza e non interviene a sostegno di tutti quei milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure, perché non hanno i soldi; una legge di bilancio - vi ricordo - dove il *super ticket* viene abolito con una cifra ridicola e, quindi, rimane.

che vediamo comparire in Assemblea, con piacere, la ministra Lorenzin, assente durante tutto il dibattito e le votazioni del disegno di legge sul biotestamento,

per le categorie professionali sanitarie. L'obiettivo è fare in modo che ci sia una regolamentazione, che era necessaria da diverso tempo e - soprattutto - che serve in modo razionale e fondamentale per la lotta all'abusivismo sanitario; di mettere in sicurezza in modo particolare la salute dei cittadini, affinché il cittadino che si rivolge a queste categorie abbia la certezza e la garanzia di una regolamentazione ben precisa. Quindi, da questo punto di vista, su questi aspetti del provvedimento noi abbiamo un giudizio convintamente positivo. Permangono le perplessità, come ho detto precedentemente, relativamente alla regolamentazione degli ordini professionali. Prendiamo atto però del fatto che la discussione di questa mattina e l'approvazione di alcuni ordini del giorno vanno nel senso di porre rimedio ad alcune manchevolezze

siccome il provvedimento è una delega al Governo e, quindi, non una legge, mi auguro che, essendo presente il Ministro della salute e i rappresentanti del Governo, nella delega si tenga conto in modo particolare degli degli impegni che sono stati assunti, perché gli ordini del giorno, che solitamente sono un contentino per ottenere l'approvazione del provvedimento, in questo caso siano un impegno preciso. Con queste motivazioni il voto di Forza Italia sarà, non convintamente, favorevole.

che il testo legislativo al nostro esame sia complesso per le tematiche che affronta. Come abbiamo visto anche nel voto, ci sono diversi gradi di gradimento

è il presupposto per regolamentare e questo è un principio che vale in tutta Europa. È così che dobbiamo leggerle, non come corse o rincorse. Certo, sarà difficile, ed è difficile

che è quella di rispondere e mettere al centro i bisogni della persona assistita, guerre non ce ne devono essere e non ce ne saranno. Mi soffermo quindi sulle altre

in quanto nel testo sono contenuti alcuni punti fondamentali per l'attività quotidiana e il futuro delle professioni sanitarie. Guardiamo con particolare interesse alla risposta che viene data ad oltre un milione di cittadini e di operatori che, giorno dopo giorno, svolgono un lavoro assolutamente proficuo nell'interesse e nella tutela della salute pubblica. Siamo molto interessati e guardiamo con positività al segnale fortissimo che viene dato alla lotta all'abusivismo sanitario, ma ci sono alcune questioni che non ci sono piaciute e che non ci hanno convinto. Tra i profili critici degli ordini segnalo, in particolare, che il testo limita in modo discriminatorio la libertà di voto degli iscritti nella loro funzione di elettori; non vengono affrontati problemi di sostanziale importanza quali il rapporto e il coordinamento con l'autorità giudiziaria nell'ambito disciplinare; l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari è affidata ad una terna di sorteggiati tra gli iscritti, senza alcuna caratteristica o qualificazione. Ritengo che sia giusto, così come previsto nella norma, separare la fase istruttoria da quella giudicatrice, ma l'istruttoria deve essere sicuramente affidata a soggetti competenti e qualificati. Altro punto critico è la costituzione di seggi diffusi negli ospedali delegando al Ministro le regole per la costituzione dei seggi stessi, senza tener conto del tema dei costi di un'operazione di questo genere e senza che la norma contenga o espliciti

moltissimo il Governo, tutto il Parlamento, le colleghe, i colleghi e gli Uffici che hanno fatto un lavoro davvero straordinario in questi lunghi anni di esame di un provvedimento storico. La ministra Lorenzin si associa. Penso che sia doveroso il ringraziamento per un lavoro senza sosta di grande qualità. *(Applausi

e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico

onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, faccio una brevissima illustrazione sulla filosofia di questo provvedimento che è rimasta inalterata e risponde a una duplice esigenza. prima è adeguare l'ordinamento italiano agli indirizzi del CIO, aumentando a tre il numero massimo dei mandati dei vertici del Comitato olimpico nazionale. La seconda è estendere tale disciplina anche agli organi di vertice delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Tale previsione si rende necessaria in quanto la normativa attuale prevede, per i presidenti federali, di poter essere rieletti dopo due mandati consecutivi a patto che ottengano il 55 per cento dei voti validi. Questo in passato ha permesso lunghissime permanenze in carica. Come già previsto nella versione del disegno di legge approvata dal Senato, la nuova disciplina si applica anche agli enti di promozione sportiva e alle strutture territoriali di CONI, federazioni sportive e discipline associate. Inoltre, essa si estende nelle stesse misure descritte anche all'intero universo paralimpico, oggetto della recente disciplina dettata dal decreto legislativo n. 43 del 2017, attuativo della riforma Madia, intervenuta mentre il presente provvedimento era in corso di esame a Montecitorio. Per tale ragione la Camera, in coerenza con la nuova disciplina organica del Cip, delle federazioni sportive e delle discipline associate paralimpiche, è intervenuta novellando il predetto decreto, come prevede l'articolo 3 del disegno di legge. Nella sostanza, tuttavia, il contenuto delle disposizioni già contenute nel testo del Senato è rimasto inalterato. Passando a un breve esame dei contenuti principali del provvedimento e delle modifiche più significative, si segnala come l'articolo 1 sia identico, disponendo che gli organi del CONI possano svolgere a regime tre mandati. Lo stesso numero massimo di mandati è previsto all'articolo 2, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 per gli organi direttivi delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, demandando la previsione agli statuti federali in coerenza con il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Questo è un passaggio comunque molto importante da prendere in considerazione. La prima novità prevista nel testo approvato alla Camera è che i medesimi statuti dovranno promuovere le pari opportunità tra uomini e donne. La seconda, di natura prettamente linguistica, ha riguardato la sostituzione della parola revisione con riduzione in materia di deleghe di voto nelle assemblee elettive. Al riguardo, conviene comunque ricordare come esse possono arrivare attualmente fino a 40. Il nuovo limite stabilito limite stabilito dalla legge, invece, è 5. La modifica più rilevante per quanto riguarda il contenuto è inerente alla disciplina transitoria per i vertici delle federazioni e degli enti di promozione sportiva attualmente in carica, prevista all'articolo 6, commi 4 e 7. Si prevede che coloro che sono in carica all'entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il nuovo limite dei tre mandati, con disposizioni che si applicano sia per l'universo dei normodotati che per quello paralimpico, ne potranno svolgere uno ulteriore e non due, come prevedeva la previgente versione della disciplina transitoria. Per i presidenti, in ogni caso sarà necessario assicurarsi il 55 per cento dei voti validi. Infine, sono stati esclusi dall'articolo 6 il CONI e il CIP.

Su questo articolo non abbiamo voluto mettere né democrazia né chiarezza per quanto riguarda il CONI e le elezioni. presentato degli emendamenti all'articolo 3 che chiedevano che non potessero ricoprire il ruolo di Presidente coloro che partecipano ad altri organi a indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Noi votiamo convintamente contro questo articolo che non è stata modificato in alcun modo e che dimostra al Paese di non voler garantire un sport

Approvando questo emendamento abbiamo uno spiraglio, un minimo spiraglio. Si chiede in questo emendamento di non poter esprimere non più di tre preferenze tra i candidati. Chi conosce il meccanismo delle votazioni sa bene che più aumenta il numero di preferenze e più è facile indirizzare i voti. Chiedo all'Aula un senso di responsabilità minimo.

Spero che almeno su questo ciascun senatore si possa rendere conto che non abbiamo consentito allo sport in Italia di avere il giusto rispetto che merita. Abbiamo riscritto il documento il documento e abbiamo voluto negare quello che si era conquistato in un primo tempo in Commissione al Senato. Spero Spero che perlomeno, per quanto riguarda la scelta che è riferita alle pari opportunità tra donne e uomini, si possa ripristinare un minimo di diritto alla

l'emendamento 6.9 si chiede che «i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati». Non abbiamo toccato i limiti, sono rimasti tre e addirittura non vogliamo che decada

le realtà che ci sono e chi chiede le tutele. Credo però che, se c'è una possibilità per dimostrare un minimo di rispetto,

per lo *sport* italiano: il limite delle cinque deleghe che possono essere rappresentate in Assemblea e, soprattutto, il fatto che il limite dei mandati vale anche per gli enti territoriali. In tali enti ci sono stati dei "condizionatori" dello *sport*, e lo sa bene il presidente Sibilia che è stato l'unico che è riuscito a commissariare la sua federazione, nel suo territorio, per un

per dire che condivido le considerazioni del senatore Ranucci. Mi sembra che il disegno di legge che stiamo approvando razionalizzi una situazione, sia frutto di una lunga riflessione e dia certezze al mondo dello sport, dopo un'attesa lunga e un *iter* molto travagliato. Quindi non è singolare che in fine di legislatura, o comunque alla fine di questa sessione che precede il Natale, si discuta questo tema, perché in Italia l'organizzazione dello sport

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali dichiaro il nostro voto contrario al provvedimento Si tratta di un'occasione colpevolmente mancata, perché lo sport italiano avrebbe avuto bisogno di un intervento sulla sua *governance* e struttura, una legge quadro che, ancora una volta, non è arrivata. E questo in base al principio sacrosanto che lo sport e la sua diffusione costituiscono una politica pubblica per eccellenza in termini di salute, di inclusione delle persone, di educazione, di formazione della personalità e anche per lo sviluppo economico. Lo sport, infatti, vale il 2 per cento medio del PIL in Europa, non solo il calcio ma l'impiantistica sportiva, l'abbigliamento, gli istruttori, i corsi, lo sport di base, con una presenza vasta e diffusa nella società che non è mai abbastanza. Tutto ciò, in Italia, caso unico in Europa, è governato dal 1942 con una delega al CONI che ha assunto lo stato di ente pubblico. Allo Stato italiano è rimasta solo una funzione di mera vigilanza statutaria.

mancano un piano e un censimento delle attività sportive del Paese; scarseggiano le campagne per la diffusione dell'attività sportiva e di uno stile di vita sano,

Questi sono i problemi che avremmo dovuto affrontare e non l'abbiamo fatto. Ci stiamo limitando a un piccolo intervento, a un mediocre intervento, che non può giustificare il nostro sostegno. *(Applausi

posso subito affermare che, dalla proposta iniziale dei colleghi Ranucci e Puglisi, oggettivamente si sono fatti notevoli passi in avanti, come anche il collega poco fa ha voluto ricordarci. Dunque, non vi è dubbio che ci si è mossi in una direzione, con una maggiore attenzione mai sufficientemente all'altezza del livello che lo sport italiano e la funzione sociale che lo sport esercita senz'altro meritano. Non vi è dubbio che parliamo oggi del Comitato olimpico. Ma l'inserimento anche del Comitato paralimpico, che nel decreto legislativo n. attenzionato come meritava già allora, ma anche i cambiamenti che si sono poi succeduti, di fatto, hanno riservato delle concrete attenzioni. Dunque, l'attività del Comitato italiano paralimpico giustamente dev'essere attenzionata ma, nello stesso tempo, deve il limite dei mandati - sostanzialmente ci si riduce a questo - è oggettivamente riduttivo parlare di esso quando si parla del significato dello sport italiano. Non vi è dubbio che il sottoscritto abbia sempre riservato delle serie perplessità serie perplessità anche nei confronti di chi, di fatto, presentandosi all'appuntamento elettorale, veniva sostenuto, eletto con un consenso assolutamente democratico. Dunque è una cosa è una cosa positiva porre dei limiti. Temo che questo, in futuro, limiterà non poco la credibilità dei nostri rappresentanti nel contesto internazionale. Pochi stanno attenzionando il ruolo e le persone straordinarie che hanno assolto e stanno assolvendo a un compito nel

Non c'è dubbio che la credibilità del nostro sistema non solo sportivo passa anche per l'inserimento nel contesto internazionale dei nostri delegati del Comitato olimpico internazionale e, più in generale, dei Presidenti delle federazioni internazionali.

una sfida alla quale ci siamo sottratti, di fronte alla quale siamo scappati, e di cui ci siamo resi prima protagonisti con la credibilità che ha lo sport italiano nel mondo, e poi ci siamo resi ridicoli con una decisione presa da qualcuno che a lei è molto caro, ma non certo a me né a noi.

ci troviamo in seconda lettura al Senato a dibattere frettolosamente di questioni importanti, stretti tra le pressioni lobbistiche del CONI e delle federazioni sportive e la necessità di occupare il tempo in attesa del ritorno della legge di bilancio. Lo sport è molto importante per i cittadini e per il Paese. Quindi, è molto importante il metodo di governo e il tempo di governo concesso a chi ricopre un ruolo apicale nel CONI e nelle tante altre associazioni che si occupano dell'organizzazione sportiva. Per questo motivo la *governance* e il ruolo del CONI e delle federazioni hanno bisogno di cambio generazionale, che con questo provvedimento non ci sarà, e purtroppo perderemo l'ennesima occasione per migliorare le nostre regole e quindi i comportamenti e i risultati.

Per quanto riguarda ciò che oggi andiamo ad approvare, temo che la quantità di denaro che muove lo sport, così come il numero altissimo grazie a tutta preferisce cooptare sempre le stesse vecchie facce e gli stessi dirigenti, che non hanno del tutto fatto del bene allo sport. E non mi accanisco sull'incredibile eliminazione della nostra Nazionale ai Mondiali di calcio. In quest'Aula, almeno una cosa, in un primo momento, era stata conquistata: il limite dei due mandati e quello a una sola delega esercitabile nel caso di voto per l'elezione dei presidenti e dei membri degli organi direttivi delle federazioni; ipotesi subito azzoppata dalla relatrice di allora, grazie a una disciplina transitoria, che ha consentito di salvare e ripescare per altri due mandati i dirigenti in carica. Ottima pesca! Peccato che i pesci siano i nostri atleti e i nostri figli! poi intervenuto il lavoro della Camera, che ha modificato in più parti il testo approvato in Senato. Faccio una carrellata sintetica, limitandomi esclusivamente a quelle che ritengo le peggiori modifiche apportate. Una volta superata la fase transitoria, è aumentato a tre il numero massimo di mandati del presidente e degli altri componenti della giunta nazionale del CONI. Per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, sempre nel numero di tre - per voi perfetto - è individuato il limite ai mandati dei Presidenti.

dei mandati esercitabili dal presidente e dagli altri componenti della giunta nazionale. E tutto ciò è fatto a vantaggio degli atleti paralimpici; ma consentitemi

il vantaggio è solo per chi vuole mantenere la carica già ricoperta, magari sperando in una forma di successione dinastica, con buona pace della democrazia. alla perla finale: i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica, che all'entrata in vigore della legge sono in carica e hanno già raggiunto il previsto limite di tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei presidenti,

Una perla, dicevo: fatta la regola, approvate anche la deroga e la proroga. Certo, sempre meglio di nessun limite, dite voi; sempre meglio una legge mal fatta, che nessuna legge. Di fatto, i tre mandati e la deroga descritta rischiano di ripristinare l'assenza del limite. E questa non è una riforma, ma è una controriforma, che prolunga il potere di chi l'ha A proposito di mancanza di limite, concludo stigmatizzando il malvezzo per cui si provano a inserire emendamenti alla legge di bilancio in un'Aula, mentre l'altra discute un intero provvedimento per due volte, dedicandovi in - quello sì - tempo, passione ed energia. Per questo ringrazio anche la relatrice Idem. Mi riferisco al fatto che alla Camera dei deputati, durante i lavori sulla legge di bilancio, dopo che era stata approvata in Senato, sono stati presentati altri emendamenti che hanno creato una distorsione nell'*iter* legislativo, senza raggiungere lo scopo. Aver proposto un emendamento per innalzare il limite dei mandati, ora limitati giustamente a due, per il solo presidente Malagò del CONI, è stata la strada originariamente prescelta. In seguito alla rivolta di tutti gli altri, è stata abbandonata la via del cosiddetto emendamento Malagò, per tornare a discutere dopo un'attività di *lobbying* serratissima da parte degli interessati, che hanno ottenuto una calendarizzazione urgente del provvedimento al Senato. Noi siamo qui a riformare il settore della dirigenza sportiva, solo perché, con un emendamento *ad personam,* è stato sollevato un putiferio, che ora dovete provare a controllare. Stiamo discutendo il provvedimento non per migliorare con serietà la legislazione - come già detto anche illustrando gli emendamenti - ma per fare gli interessi di chi è sempre stato al potere nel mondo dello sport.

per il principio dei due mandati, scaduti i quali il comando e la responsabilità passano a nuove persone motivate, capaci ed entusiaste. Nel frattempo, però, alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi per la stipula di contratti professionistici: un'altra casta, sotto la supervisione del CONI, che dovrebbe occuparsi solo delle Olimpiadi. E il Movimento 5 Stelle ritiene che quello sia il suo ruolo. Ricordate che ho detto che lo sport è importante per la quantità di denaro circolante? Ecco la prova. Il CONI sarà fondamentale, perché dovrà adottare il regolamento che stabilisce l'incompatibilità e le sanzioni sportive. Io credo che ce ne sia abbastanza per capire perché la nostra iniziativa politica è avversata da tutte politica è avversata da tutte le forze politiche, abbracciate in un fascio unico fatto di maggioranza e opposizione, unite a favore del mantenimento in carica dell'attuale dirigenza sportiva. Questo non è lo sport che vogliamo noi, né i cittadini e quanti lavorano con amore e passione, dedizione e professionalità nel campo dello sport. Per loro c'è solo onore.

poiché questa è l'ultima volta che prendo la parola in Assemblea in questa legislatura, colgo l'occasione per ringraziare la struttura burocratica del Senato per il supporto che ha dato a me e a i tutti i miei colleghi e colleghe per quattro anni e nove mesi. Grazie infinite. A me, che ero alla prima legislatura, avete consentito di lavorare nel miglior modo possibile.

Quando si è pensato che fosse opportuno porre un limite di mandati, si è cercato di procedere con una certa razionalità e tenendo conto della realtà.

Non inventiamo nulla: facciamo qualcosa che all'estero ci hanno dimostrato essere efficiente. Nell'ambito dello sport e nel mondo non esiste un organismo che abbia un numero di mandati inferiore a tre. Quasi tutte le federazioni sportive all'estero non hanno numero di mandati. Per quanto riguarda le norme transitorie, le norme transitorie, sono state studiate in modo tale da consentire che un'organizzazione, che con i suoi pregi e i suoi grandi difetti è comunque frutto di un'esperienza di cento anni, si cambi, ma senza una rivoluzione che comporterebbe un grande stravolgimento o un mondo che nel 99 per cento dei casi è di dilettanti. Mi sembrano norme di buon senso che consentono di avere un rinnovamento; fra sette anni il mondo sportivo sarà completamente rinnovato,

la Camera non ha toccato il provvedimento nella sostanza, introducendo norme di buon senso e valide per quanto riguarda la parità di genere e l'esaltazione del ruolo delle donne; anche questo senza rivoluzione, ma con un riformismo corretto. Per questa ragione voglio ringraziare la relatrice Idem, che ha messo passione, e il senatore Ranucci, che aveva presentato insieme alla senatrice Puglisi, il disegno di legge parlamentare dal quale siamo partiti. Penso che il Parlamento abbia fatto un lavoro positivo. Anche lo stimolo che è arrivato dalla senatrice Blundo,

e riconoscere la funzione sociale, formativa e di crescita del nostro Paese che esso ha avuto nei decenni trascorsi e che potrà avere sopratutto nel futuro.

Carraro. L'idea fu lanciata dal senatore Ranucci e dalla senatrice Puglisi con il loro disegno di legge perché, nel rispetto totale dell'autonomia dello sport, potevamo dare un segno di modernità, riportando nello sport delle esigenze rivelatesi rivelatesi importanti anche nel mondo della politica e delle istituzioni; l'esigenza di rinnovare col tempo una classe digerente, senza ledere l'autonomia dello sport e metterlo in difficoltà. Le federazioni sportive sono certo importanti, così come sono importanti tutte le organizzazioni

sono amareggiato solo di una questione importante. Durante quelle audizioni noi ascoltammo anche la signora sindaco Raggi per chiedere garanzie, per dare supporto e fare squadra, perché di fronte a noi avevamo un'occasione importante per il nostro Paese, quella delle Olimpiadi del 2024 a Roma. Abbiamo chiesto questa collaborazione, ci siamo resi disponibili - lo ha fatto il Governo e lo ha fatto tutto il Parlamento - proprio in occasione di quella audizione. Abbiamo trovato sordità; secondo me abbiamo trovato anche cecità. avviso, avete fatto degli errori e questo è stato un errore grave. di pensare che con quella decisione voi abbiate lavorato contro il nostro Paese e contro la città di Roma.

hanno parlato tutti; adesso ha diritto di parlare anche il senatore Marcucci.

Mi permetto ancora di dire che noi del Gruppo del Partito Democratico siamo felici e orgogliosi di arrivare alla votazione di oggi.

ci è portato. MARCUCCI *(PD)*. Mi permetto di concludere sottolineando l'orgoglio del Gruppo del Partito Democratico nell'aver lavorato per rafforzare lo sport in questo Paese e averlo modernizzato. Questo provvedimento va in questa direzione. direzione. Concludo con l'augurio di buon lavoro alle federazioni, al Comitato olimpico e a tutti gli sportivi italiani. Grazie.

trasmessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari.

trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma - nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale

il Gruppo Articolo 1-MDP voterà contro, essenzialmente e molto in sintesi per due ordini di ragioni. Innanzitutto, riteniamo che un delitto quale quello di vilipendio, così come configurato, sia un retaggio antistorico. Va affrontata la questione della rispettabilità e della dignità, in questo caso delle Assemblee parlamentari, in altra maniera: la critica va comunque consentita. Non vogliamo intervenire certamente nella vicenda che ha visto in più occasioni contrapposti il senatore Albertini e il dottor Robledo. Ci limitiamo a una considerazione di carattere giuridico-costituzionale ed al codice penale. Inoltre, riteniamo che il Parlamento, più che entrare in vicende giudiziarie penali di questo genere, dovrebbe difendere la propria onorabilità con un lavoro costante, preciso e trasparente, tenendo sempre presenti i criteri di dignità previsti dalla nostra Costituzione. Per questi motivi, voteremo contro

l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti di chi si rende potenzialmente responsabile del reato di vilipendio alla Repubblica e alle Assemblee legislative (reato previsto dall'articolo 290 del codice penale) prevede una proposta favorevole. Per la prima volta, cioè, il Senato si appresterebbe, qualora venisse approvata la proposta della Giunta, a far sì che si proceda giudizialmente per sanzionare, sia pur con una pena di natura pecuniaria, chi avrebbe vilipeso l'Assemblea legislativa. La vicenda del dottor Robledo notoriamente - non è un segreto - si inserisce nell'ambito di un contrasto annoso tra un membro di quest'Assemblea e il predetto magistrato.

di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica, che ha visto una nostra iniziativa legislativa volta ad abrogare quella norma, addirittura retaggio di epoca monarchica e poi riportata in ambito repubblicano dal codice penale del periodo fascista,

come anche richiamato nello stesso documento, riteniamo che il prestigio, l'onorabilità e la rispettabilità degli organismi costituzionali e della stessa Repubblica debbano essere guadagnati sul campo

Non sarò certo io a voler aggiungere il carico su quanto nella percezione, talvolta anche distorta (non dico di no), dei *media* e dei *social* questa impressione sia completamente perduta, perché vi è una sensazione di sfiducia e talora anche di disprezzo per questi organismi costituzionali. Tuttavia, questo rispetto dobbiamo guadagnarcelo sul campo e non arroccandoci o dando anche la sola impressione di arroccarci dietro a quello che appare uno scudo anacronistico del punire chi critica, magari anche con violenza ma verbalmente (ovviamente parliamo di violenza verbale e giammai di tipo fisico o fattuale). Crediamo che questo tipo di atteggiamento, tanto più perché costituirebbe un un capovolgimento di 180 gradi dell'orientamento avuto finora dalla Giunta e dal Senato, sarebbe un fatto gravissimo che, anziché andare verso l'intenzione annunciata, si riverbererebbe contro il rispetto degli organi costituzionali, Senato compreso.

che, quand'anche non si condividesse il punto di vista che sto cercando di esporre, nelle frasi del dottor Robledo (riportate a pagina 2 del documento), vedrete che le sue parole sono di forte critica, certamente sgradevole, censurabile, possiamo anche dire inaccettabile, ma rimangono comunque delle opinioni, tutelate dall'articolo 21 della Costituzione. Il riferimento è alla Giunta delle immunità parlamentari

Qui, il dottor Robledo non attacca il Senato in quanto tale, bensì un organismo, in questo caso la Giunta delle immunità. Se apriamo il varco dell'autorizzazione a procedere per reato di vilipendio

Dove andremo a finire? E io dico, in questo caso: dov'è la voce di quei garantisti, dei senatori Buemi e di chi, dall'altra parte dell'emiciclo,

(Mi riferisco al garantismo che è peloso, non ai corpi dei senatori che esprimono tali posizioni). *(Commenti dal Gruppo PD).* Quello che sto dicendo avrà maggiore consistenza quando esamineremo l'altro documento, relativo al medesimo reato, cioè l'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Angelico, direttore amministrativo della Procura di Catania, che ha osato pubblicare un *post*, la cui offensività vi invito a giudicare (anzi lo faremo quando esamineremo

caso si vuole aprire un varco di punibilità da parte del Palazzo del Senato, e più in generale del Parlamento, che si sente offeso da un *post*, la cui offensività è nulla rispetto a quanto purtroppo leggiamo ogni giorno, così cadendo nella trappola

stiamo cambiando in maniera così radicale questo orientamento? Ci rendiamo conto che il risultato finale non sarà una tutela delle istituzioni, ma ancor più il loro disprezzo apparente,

veramente un segnale che varrebbe più di cento di questi documenti di Giunta, che vorrebbero nominalmente tutelare l'immagine del Parlamento. Per questi motivi, si comprende bene che il voto

perché troppe volte accade che pubblici ufficiali si lascino andare ad atteggiamenti di oltraggio a organi costituzionali e organi dello Stato in generale. In questo caso è ancora più grave che questo atteggiamento sia stato assunto da un cittadino, da un pubblico funzionario dello Stato di grado elevato, che è assolutamente in possesso degli strumenti per valutare qual è la portata del proprio atteggiamento e delle proprie affermazioni. Qui non si tratta di un cittadino normale, non acculturato rispetto alle problematiche del nostro sofisticato sistema giuridico penale: si tratta di un magistrato,

nei confronti dello Stato e dei suoi organi, si assumano atteggiamenti delegittimatori di questo tipo. La Giunta delle elezioni nell'assumere certi provvedimenti, erano nella pienezza del diritto costituzionale e nella legittimità delle proprie posizioni e quindi non può essere consentito a nessuno di mettere in discussione l'onorabilità

in effetti alcune cose vanno precisate. Intanto, si veda la giurisprudenza, o meglio la consuetudine della Giunta degli anni passati, per altro risalenti. le ultime decisioni sono state nel senso di negare l'autorizzazione a procedere, ma ad una migliore ricerca e ad un approfondimento è risultato che nel passato è stata più volte e reiteratamente concessa l'autorizzazione a procedere per casi analoghi a quelli che ci occupano.

che ha poi confermato la decisione assunta dalla Giunta. Si tratta di un attacco assolutamente duro e veemente, probabilmente perché egli si è sentito colpito nella sua persona.

«Non possono sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti». Basterebbe già questo per capire di che cosa stiamo parlando e quali sono le accuse che sono state rivolte all'Assemblea. Concordo molto

dottor Robledo nei confronti dell'Assemblea parlamentare, stiamo semplicemente valutando se dobbiamo concedere l'autorizzazione oppure no. Il giudizio su questi fatti spetterà unicamente alla magistratura. Forse dovremmo provare ad avere più rispetto reciproco delle istituzioni, e bene ha fatto il senatore Buemi a ricordare che chi ha parlato non è uno qualsiasi, ma un magistrato e da magistrato dovrebbe avere fiducia nelle istituzioni, di cui lui stesso fa parte. Bottici).* Noi dobbiamo semplicemente limitarci a concedere l'autorizzazione a procedere, ovvero quella condizione di procedibilità senza cui non si potrebbe andare avanti nel procedimento e non si potrà mai sapere chi abbia ragione. In questo caso, ripeto, la giurisprudenza costante dice che quando la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo il destinatario al disprezzo e alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa. Basti dire che ci ha accusato di aver attuato un voto di scambio, ci ha accusato, in buona sostanza, di aver commesso un reato. Se non ci sono le condizioni in questo caso per concedere l'autorizzazione, allora non so quando vi siano; allora dovremmo avere il coraggio di di abolire direttamente l'articolo 290 e dimenticarlo. Possiamo occuparci di questo, ma vigente questo codice penale, vigente il nostro sistema, noi abbiamo il dovere di difendere le istituzioni. Si ricordi che le decisioni di cui si è parlato sono molto risalenti nel tempo, molto risalenti nel tempo, al punto che non esistevano, in quel periodo, i *social*. Oggi siamo presi di mira nella quotidianità del nostro operato e anche quando operiamo bene, c'è sempre qualcuno che ci insulta. Forse dovremmo cercare di stare un po' più uniti nella difesa di queste istituzioni, perché credo sia un nostro dovere per il giuramento che abbiamo prestato alla Costituzione, perché questi sono diritti che sono contenuti nella Costituzione e in questo senso dovremmo essere un po' più uniti e difenderla, lasciando ad ognuno il proprio compito. Il giudizio spetta alla magistratura di fronte alla quale, anche in altre circostanze, ci siamo inchinati e siamo sempre pronti e disponibili ad inchinarci rispetto al loro operato. Ma - vivaddio - svolgiamo i nostri compiti, perché credo che l'autorevolezza la guadagniamo anche espletando onestamente e giustamente i nostri compiti.

mi ha incuriosito molto l'intervento del senatore Buccarella e conseguentemente sono andato a leggere gli atti di questa delibera della Giunta. Vorrei molto rapidamente dire pochissime cose. In primo luogo, siete tutti contrari all'esistenza del reato di vilipendio: mi spiegate la ragione per la quale avete osteggiato la modifica del reato di vilipendio in quest'Aula e, successivamente, quella modifica che era stata varata in quest'Aula è stata poi bloccata alla Camera? Forse perché in quel caso il reato di vilipendio trovava come imputato Francesco Storace? Secondo punto: vede, senatore Buccarella, lei si chiedeva dove sono i garantisti, il senatore Buemi e quelli di questa parte dell'emiciclo. Sa, senatore Buccarella, riflettevo: voi avete sempre votato favorevolmente alle richieste di un magistrato;

l'autorità giudiziaria ha la possibilità di sollevare conflitto e, sulla base del conflitto, la Corte costituzionale si pronuncerà. Vede, senatore Buccarella, nel caso di specie, l'assenza dell'autorizzazione da parte del Senato comporterebbe la chiusura di quelle indagini cui il procuratore di Catania sembra interessato, indagini che il procuratore di Catania ritiene utili ravvisando quantomeno quel minimo di indizi che gli impedisce l'archiviazione immediata. Allora capirà, senatore Buccarella, che io sono interessato a votare questa autorizzazione per una ragione molto semplice: il dottor Robledo ha accusato il Senato, nella sua conformazione plenaria e nella sua conformazione di Giunta, del reato di abuso in atti d'ufficio e del reato di voto di scambio. Io non voglio bloccare le indagini dell'autorità giudiziaria, voglio capire se questo è realmente accaduto perché il dottor Robledo si dovrà necessariamente difendere e ci spiegherà sulla base di quali elementi ha fatto delle affermazioni così gravi. Siccome io faccio parte di questo Senato, ho tutto l'interesse che, sia pure *pro quota*, quella *pro quota* di immagine che mi riguarda sia affrontata da quell'autorità giudiziaria nei cui confronti voi e tutti noi manifestiamo rispetto. Ho l'impressione che voi manifestiate un rispetto formale a senso alternato.

anch'io mi ero aggiunta alle persone che hanno manifestato perplessità sul reato di vilipendio, ma fino a che il reato di vilipendio esiste ed è presente nel nostro ordinamento,

sulla colpevolezza o innocenza, trattandosi semplicemente di una condizione di procedibilità, sarà doverosamente espresso dall'unico potere dello Stato cui ciò è riconosciuto, cioè la magistratura.

malgrado la Giunta delle elezioni avesse deciso, con il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle, che sarei dovuto andare sotto processo per una dichiarazione che avevo fatto all'esterno del Parlamento

lo facciamo convintamente. Chi vi parla, nel lontano 1999, da umile e semplice sindaco di Aulla, ha avuto un fascicolo aperto per vilipendio alla Costituzione. Il reato che aveva commesso era stato denunciato da 76 deputati dell'allora Partito Democratico, ex Partito Comunista, perché come membro del Consiglio comunale avevo osato dare la cittadinanza onoraria a Bettino Craxi e portargliela in vita. Ovviamente poi il fascicolo è stato chiuso, perché il Governo D'Alema, di allora, aveva offerto i funerali di Stato e, a quel punto, il procuratore, pur avendo aperto il fascicolo di vilipendio,

che permette di mettere su Facebook un'immagine raffigurante il dito medio alzato collegato alla bandiera italiana e di scrivere «un caro saluto ai nostri amati parlamentari da parte di tutti noi italiani», sostituendosi quindi ad facente parte di un'istituzione costituzionalmente codificata.

la dottoressa Sabrina Angelico non è un magistrato, è un dirigente amministrativo. Vorrei sottoporre questa particolare vicenda all'attenzione del Senato, perché non vorrei che si superasse il senso del ridicolo. Premetto una questione di carattere giuridico. L'autorizzazione a procedere della quale stiamo dibattendo è una condizione di procedibilità così come, *mutatis mutandis*, la querela. per capirci: cos'è la querela, ad esempio, per il delitto di diffamazione? Significa che la parte che si ritiene offesa effettua una valutazione giuridica, di fatto complessiva, al fine di chiedere al giudice di procedere per la punizione del presunto responsabile. Questa è la situazione processuale penale. A noi viene chiesto se, in questa situazione, come nella precedente, il Senato, in quanto parte offesa, ritenga di dover chiedere di procedere per la punizione. Sono quindi schemi falsi quelli per cui si dice che valutiamo solo la procedibilità, senza entrare nel merito, perché il Senato, quando autorizza questa richiesta, chiede il processo e la punizione della persona che ritiene colpevole, ovviamente e giustamente in presenza delle prove. Questo quindi è il dato di carattere rituale processuale. Parlavo di senso del ridicolo. Rischiamo, come Senato e come Parlamento, di essere inondati di messaggi e *post* sui *social network*. Ricordo qual è la situazione: la presenza di un dito medio alzato e di una frase - e avremo sentito molto peggio - che viene ritenuta vilipendiosa, diffamatoria: «un caro saluto ai nostri amati parlamentari, da parte di tutti noi italiani», con quella raffigurazione. Provate a immaginare cosa potrà succedere oggi o domani: il Senato rischia di essere inondato di migliaia, anzi di milioni di queste dita alzate per una vicenda del genere. Per questo dico non superiamo il senso del ridicolo torniamo a valutare quello che è questo delitto di vilipendio da noi sempre considerato fuori dalla storia e riteniamo se sia il caso di impegnarci in un processo penale per queste vicende. Presidente, in sede di Giunta avevo manifestato qualche perplessità rispetto a un provvedimento così importante, come l'autorizzazione a procedere, nei confronti di questa pubblica funzionaria del Ministero della giustizia. Mi hanno convinto però i colleghi rispetto a un punto: qui non si tratta, come anche nel caso precedente, di un cittadino qualsiasi. Si tratta di pubblici funzionari con responsabilità elevate: nel caso precedente, di un magistrato; in questo caso, della dirigente di un ufficio giudiziario (se non ricordo male, quello di Catania)

La capacità di valutare i fatti e i comportamenti, nonché la loro rilevanza rispetto al codice penale, è normale per un pubblico funzionario che opera nel settore della giustizia. Quindi, c'è la consapevolezza dell'atto. Si tratta pur sempre di un dito medio alzato verso il cielo (cosa che succede per milioni di casi in rete), ma la non è la stessa di quella di un cittadino qualsiasi che, dopo una giornata di lavoro stressante, si mette alla tastiera e alza il dito verso il cielo con qualche commento sgradevole. Qui c'è un problema di cultura

in questo caso specifico, si sono assunti la responsabilità di affermare cose sgradevoli a nome del popolo italiano e, in questo caso credo che, come ha giustamente ricordato prima il collega Cucca, noi dobbiamo arrivare in una sede in cui cominciano a rimettere i puntini sulle i nella maniera opportuna. C'è un'autorità giudiziaria che deve esprimersi su determinati atti che è chiamata a giudicare. Se si pone un problema di

Vedo anche l'attuale capo del partito, a cui il senatore Palma credo appartenga ancora, Berlusconi. Anche lì vedo fotografie e ritratti col dito medio.

veniva giustamente ricordato, equivale di fatto a una sorta di querela. È come se noi, in quanto Senato, ci ritenessimo offesi dal post di una cittadina siciliana e volessimo querelarla. Qui - ribadisco - apriremmo un varco che ci porterà al triste e *cupio dissolvi* del principio di responsabilità, di rispetto e di onorabilità di un'Istituzione parlamentare. Per carità, non cadiamo in questa trappola, né tanto meno abbiamo intenzione di cadere nella trappola del presunto contrasto tra magistratura e politica, che qui non c'entra assolutamente nulla e voglio che questo sia chiaro, anche in replica a ciò che è stato oggetto dell'intervento del senatore Palma. Per questo motivo annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle al documento in questione.

poi le festività e il ritorno a casa. Stiamo però attenti a non commettere un errore imperdonabile. Non si può essere così attenti e così preoccupati della sorte di qualunque parlamentare per il quale sia stata chiesta un'autorizzazione e poi essere così leggeri quando si tratta di perseguire una persona che è fuori dal Parlamento. Come sapete, sono tra quelli che ha difeso strenuamente la Costituzione dato che quello era il contesto, ho difeso anche la permanenza di questo Senato e ne sono, tutto sommato, orgoglioso. Stiamo attenti però a non eccedere. La polemica contro la casta è anche distorcente, ma esprime una profonda delusione di una parte del Paese, perché la politica non riesce a rispondere alle domande reali della cittadinanza. Gli atteggiamenti che ho sentito oggi in Assemblea anche da persone, da senatori, dai quali non me lo sarei aspettato, sono veramente atteggiamenti di casta. Per favore, fermiamoci un momento prima di fare una sciocchezza sotto Natale.

opportuno avere una certa manica larga da parte del Senato nei confronti di cittadini che, esprimendo le loro opinioni, possono farlo in modo magari anche

e magari possibilmente garbata contrarietà alla cosiddetta classe politica (entità che non ritengo esista), ma ad un attacco alle istituzioni in quanto tali.

la magistratura deve godere del prestigio e del rispetto che le è dovuto.

al Parlamento in quanto tale. Il Parlamento, dovremmo ricordarcelo almeno quando ci siamo dentro, non è un orpello, perché in tutti i Paesi democratici, dove c'è democrazia e libertà, c'è il Parlamento: ci sono Paesi che hanno il Parlamento e non hanno democrazia e libertà perché è un Parlamento finto, ma non esiste un Paese che abbia democrazia e libertà che non abbia il Parlamento. Pertanto, quando un impiegato dello Stato, per di più in in un ufficio di particolare delicatezza, attua un comportamento di questo genere, noi abbiamo il dovere di chiedere questo e non perché ne facciamo parte - dimentichiamo di farne parte

la possibilità, ma il dovere di difendere il Parlamento. Settanta o ottant'anni fa in questo Paese sono morte delle persone, degli italiani e anche degli stranieri, per salvare la democrazia e la libertà. A loro è costato parecchio caro; a noi costa un voto

non capisco perché ci sia poi chi vuole fare delle leggi particolari nei confronti di chi in qualche modo si richiama al fascismo. È più pericolosa una bottiglia con la faccia del duce sull'etichetta o qualcuno che dice che il Parlamento va insultato perché è il Parlamento?

Ricordiamo che la democrazia è importante e non si può attaccare in quanto tale. C'è tutto il diritto di criticare i singoli atti, persino il Parlamento nel suo insieme, ma non perché è Parlamento, mentre questo è ciò che ha fatto questa signora. brevemente soltanto per ribadire ancora una volta che questa Assemblea non ipotizza assolutamente nulla. Chi ha ipotizzato la sussistenza di un reato eventualmente è il magistrato e noi stiamo semplicemente

nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito, trasmessa dal tribunale di Torino - sesta sezione penale. La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento

Anche qui, e magari lo ripeterò come richiamo al prossimo documento, valgono le considerazioni svolte in precedenza. Al di là delle legittime richieste e aspettative di ogni singolo senatore, che vuole vuole applicare un istituto che noi riconosciamo e rispettiamo, quello della insindacabilità per i voti e le opinioni espressi anche *extra moenia*, l'impressione è che molto spesso ci si faccia scudo in maniera strumentale per esercitare la propria libertà di opinione, che deve essere sempre riconosciuta, anche al di là di quanto sarebbe legittimo fare nell'espletamento di un mandato parlamentare condotto secondo criteri di equilibrio, di pacatezza, ma anche di determinazione contro alcune iniziative, come nel caso di specie. Pertanto, il voto del nostro

costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. **È approvata.**

nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Paola Taverna, trasmessa dal tribunale di Roma - sezione del giudice per le indagini preliminari». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Paola Taverna non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

non deve essere affrontato in maniera tale da discriminare tra maggioranza e opposizione, tra simpatia e antipatie. Con il Gruppo del Movimento 5 Stelle, come è noto, io non ho mai avuto rapporti se non conflittuali.

mafia a Roma, di mafia Capitale, le valutazioni sulle passate amministrazioni o sui passati sindaci erano largamente coperti da interrogazioni, interpellanze e interventi fatti in Aula, esattamente come quelli del senatore Stefano Esposito o di altri colleghi per i quali giustamente è stato richiamato questo principio, ho detto che anche alla senatrice Taverna andava applicata la stessa regola che era stata applicata in questa legislatura a tutti i colleghi. Ha esercitato un suo diritto esprimendo un'opinione che aveva già espresso chiaramente in Parlamento, quindi sinceramente non ho capito perché, con i due voti di astensione del Movimento 5 Stelle, la proposta (che ha avuto sei voti favorevoli,

e quello di cui stiamo discutendo in questo momento, che riguarda la senatrice Paola Taverna. È vero che il senatore Giovanardi, quando era relatore e durante i lavori della Giunta, aveva proposto di dichiarare la sussistenza della insindacabilità ed è altrettanto vero che questa proposta non aveva raggiunto la maggioranza semplicemente per un gioco di votazioni a favore, contro e di astensione, che ha determinato una maggioranza spuria, sostanzialmente quella che ha portato a non ritenere opinioni opinioni espresse nell'ambito delle funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, quelle della senatrice Taverna. Io credo invece che queste dichiarazioni siano ampiamente coperte dall'articolo 68 della Costituzione, proprio perché fanno riferimento a fatti storici, processuali, politici e sociali di cui si è ampiamente discusso non soltanto nel Paese, non soltanto nelle aule giudiziarie, ma anche in questo Senato, da parte della stessa senatrice Taverna.

Io non so per quale motivo dovrebbe finire sotto processo per dichiarazioni dichiarazioni che credo gran parte di questo Senato condivida e quindi voteremo contro questa proposta del relatore di ritenere non corrispondenti alle funzioni parlamentari le dichiarazioni della senatrice Taverna.

corre il rischio di dover affrontare, ben consapevole della strumentalizzazione in malafede che ieri, oggi e domani, nella comunicazione pubblica quando si vuole attaccare una forza politica. Questo forse sarebbe normale, se fossimo in un Paese normale e con un'informazione normale.

ha prodotto la documentazione relativa alla quantità di interventi e interrogazioni che ha presentato su Mafia capitale, ha rappresentato la situazione e si è richiamata alla giurisprudenza e alle valutazioni della Giunta, senza voler condizionare

ci siamo astenuti, senza sapere ancora quale sarebbe stato l'esito finale. L'esito è stato quello che conosciamo tutti e che ha fatto sì che la prima proposta della Giunta fosse rigettata e ora, con la firma del senatore Cucca, viene riproposta come non riconoscimento della Noi semplicemente affrontiamo questa tematica,

dalle nostre posizioni, che - lo ribadisco - riconoscono e rispettano l'istituto dell'insindacabilità. Con riferimento alla proposta della Giunta il nostro voto sarà favorevole, perché la senatrice Taverna in questo caso non ha assolutamente nulla da temere da un eventuale procedimento penale, perché

che i grillini rinunciano al ruolo di parlamentare e a una prerogativa che è stata ideata secondo rispettabilissimi criteri che devono garantire la libertà di azione politica di qualsiasi parlamentare e di qualsiasi forza politica, ma proprio per far risaltare la grande ipocrisia

è suo diritto e l'Assemblea si pronuncerà. Nel caso del documento in esame il voto del Movimento 5 Stelle sarà a favore della proposta della Giunta per mandare un segnale che abbiamo cercato di esprimere in cinque anni di legislatura e, da ultimo, in questa mattinata di votazioni, avendo avendo richiamato il principio che il rispetto, l'onorabilità e il prestigio delle istituzioni repubblicane e di rango costituzionale, comprese quelle dei singoli parlamentari, vanno conquistati non utilizzando strumentalmente, a proprio favore o a danno di altri componenti di altre forze politiche, politiche, gli strumenti parlamentari di garanzia della libertà di opinione e di azione politica dei parlamentari. Con la massima coerenza che possiamo esprimere, senza alcuna ingenuità, ma senza ipocrisia, voteremo a favore del documento in

apprezzo il fatto che il Movimento 5 Stelle voterà a favore della proposta della Giunta, anche se ricordo ai senatori del Movimento 5 Stelle che il voto che andiamo ad esprimere in questo momento concerne la valutazione dei fatti e, in ragione della valutazione dei fatti, la valutazione sull'esistenza o meno della cosiddetta insindacabilità. Male sarebbe distorcere questo voto a uno scopo completamente diverso, che sarebbe quello, come ha detto chiaramente il senatore Buccarella, di non esporsi ad una polemica strumentale con riferimento alle loro posizioni sui privilegi, sulla casta e quant' altro. Esattamente lo stesso sarebbe se ciascuno di noi dovesse votare non con riferimento ai fatti, ma con riferimento alla posizione politica che il soggetto interessato esprime in quest'Aula.

la senatrice Taverna trattò il tema nel 2014 e nel 2015, ma che verrebbe meno il requisito della contestualità in quanto il *post* incriminato sarebbe del 2017. Questo pone un primo problema e cioè, fino a quando le dichiarazioni rese in questa Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzione, possono scriminare il soggetto per le dichiarazioni rese successivamente e credo che questo sia davvero difficile da determinare. Ancora, quello che mi lascia molto perplesso nella relazione è che, anche volendo aderire alla non contestualità temporale delle dichiarazioni, forse la Giunta avrebbe dovuto soffermare la propria attenzione sul fatto che il *post* è assolutamente contestuale al procedimento penale in corso su mafia capitale e alle dichiarazioni di Buzzi, il che evidentemente il che evidentemente contestualizza, indipendentemente dalle originarie dichiarazioni, quanto la senatrice Taverna ha inteso formulare nel suo *post*. di una motivazione estremamente pericolosa, secondo me non sintonica con la giurisprudenza ed è questa la ragione per la quale personalmente voterò contro la proposta della Giunta.

stata raggiunta da un procedimento. Ho saputo di avere un procedimento in corso, grazie alla Giunta, alla quale la Procura di Roma si è rivolta direttamente, prima di informare me, per sapere se il caso in questione ricadesse o meno sotto il profilo dell'insindacabilità. Ho fornito alla Giunta esclusivamente quanto mi veniva richiesto ovvero se, durante la mia attività parlamentare, avessi trattato il caso incriminato. Ricordo che

tanto se ne è parlato, non ho minimamente condizionato la Giunta dichiarando di avvalermi o meno di tale facoltà. Ho detto che riconosco un organo competente che saprà valutare in piena libertà quale sia la mia situazione. vi tolgo dall'imbarazzo, ringraziando - devo dire - l'onestà intellettuale di una parte di questa Assemblea e deprecando in maniera vergognosa quanto state dimostrando, facendo un discrimine esclusivamente per per appartenenza politica o forse esclusivamente perché non vi sono sufficientemente simpatica *(Applausi dal Gruppo M5S)* di fare una valutazione totalmente avulsa da qualunque logica con la quale giudicate i vostri pari, nei miei confronti e nei vostri. Ma ben venga questa differenza. Che rimanga chiara anche cittadini. Ringrazio tutti e con questo vi auguro buon Natale. simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Paola Taverna non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione)*.

L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, grazie a tutta La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento

processati come tutti i cittadini, di più, possono essere arrestati. Ahimè, ho fatto l'altro giorno il caso del nostro collega che da sedici mesi è in carcere senza che la magistratura abbia ancora deciso se ciò sia legittimo. Al parlamentare è rimasto uno scudo,

quindi se i parlamentari vengono qui semplicemente per curare i loro interessi, questa non è la funzione del parlamentare. Il senatore Stefano Esposito si batte in prima linea, in una situazione limacciosa e difficile, ha come arma quella della parola per difendere le sue posizioni, ed è oggetto di ripetute denunce. La riflessione che ho fatto mille volte

chi è che paga le spese processuali? Chi paga le preoccupazioni della famiglia? Chi non rischia di essere paralizzato nella sua attività parlamentare proprio dalla minaccia di essere continuamente sotto processo? Noi stiamo parlando della possibilità di essere liberi di fare i parlamentari, di esporci quando i cittadini non si possono esporre. Se questo coraggio che i parlamentari - o alcuni di essi - hanno di sostenere cause difficili, di scontrarsi con ambienti limacciosi, addirittura non trova la copertura dell'articolo 68 e i parlamentari devono essere sotto processo continuo e quindi passare la loro vita nei tribunali per difendersi per aver avuto il coraggio di fare delle denunce pubbliche, è chiaro che la funzione parlamentare sarebbe totalmente svuotata. Non comprendendo la posizione del PD nella votazione precedente né quella del Movimento 5 Stelle, richiamo ancora una volta i colleghi sulla necessità di salvaguardare l'unica prerogativa che noi abbiamo: i magistrati ci possono arrestare,

- Governi centristi di centrosinistra hanno sempre coperto i parlamentari della sinistra, anche quando erano accusati di reati comuni contro l'ordine pubblico perché hanno fatto sempre prevalere

Il Senato non è in numero legale.

di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del tribunale di Verona in relazione a un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco. Non risultando ancora depositata la relativa relazione, l'esame della proposta è rinviato ad altra seduta.

riprenderemo la seduta alle ore 17,30 per prendere atto dell'avvenuta trasmissione della legge di bilancio e avviare la conseguente procedura presso le Commissioni e presso l'Aula. La seduta è sospesa. *(La seduta,

grazie a tutta Vittorio Zizza hanno dichiarato di costituire il Gruppo parlamentare denominato «Noi con l'Italia» e di aver attribuito la carica di Presidente del Gruppo al senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio e di Vice Presidente alla senatrice Patrizia Bisinella. Bisinella. Pertanto i senatori Bellot, Bisinella e Munerato cessano di appartenere al Gruppo Misto e i senatori Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio e Zizza cessano di appartenere al Gruppo GAL.

una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, comunico che la Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge recante: «Bilancio di previsione

io non c'entro niente. Il provvedimento è stato deferito alla 5a Commissione permanente in sede referente e per il parere a tutte le altre Commissioni, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi immediatamente. I rapporti alla Commissione bilancio dovranno essere trasmessi in tempo utile affinché questa possa riferire all'Assemblea nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo che è immediatamente convocata. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà all'esito della Conferenza dei Capigruppo, che stabilirà i tempi per il prosieguo

la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio, che sono così stabiliti. I rapporti delle Commissioni in sede consultiva dovranno essere presentati alla 5ª Commissione permanente in tempo utile affinché questa possa riferire all'Assemblea a partire dalle ore 9 di domani mattina. mattina. Gli emendamenti per l'esame in Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre i seguenti punti già previsti dal calendario vigente: elezione dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, il documento della Giunta delle elezioni sul conflitto di attribuzione riguardante un procedimento penale nei confronti della senatrice Bonfrisco, i disegni di legge in materia di cittadinanza e sulla prevenzione dell'estremismo violento jihadista.

Signor Presidente, parimenti al mio collega Tosato, chiedo anch'io di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Calderoli sul disegno di legge in materia di cittadinanza. PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

le chiedo, cortesemente, se il Senato può essere messo in grado di valutare le eventuali liste dei candidati, esaminando anche i *curricula* degli stessi. PRESIDENTE.

Considerato che non vi è stata la votazione alla Camera dei deputati proprio in assenza di queste liste, sarebbe pura follia - ritengo - votare in una Camera e non in un'altra. Il mio è un auspicio. se non c'è massima condivisione fra i vari Gruppi parlamentari e fra Camera e Senato, io ritengo non opportuno procedere con questa votazione.

grazie a tutta